Secondo il Regolamento della Camera, Presidente, questo avrebbe comportato una riapertura dei termini. Mi si dice che il Regolamento del Senato è diverso. Signor Presidente,vorrei allora capire se il Governo, che ha sicuramente diritto di chiedere la parola e di intervenire quando vuole,

secondo la richiesta di votazione per parti separate avanzata dal senatore Palma, sul quale il rappresentante del Governo ha invitato il proponente al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

e in particolar modo mi rivolgo a quel Gruppo neocostituito che, prima della chiusura dei lavori, ha annunciato l'eventuale astensione su questo articolo e su queste sue parti.

Conosciamo tutti quell'efferato delitto; forse poche persone conoscono attentamente la storia di questo Romulus Mailat, un romeno, un cittadino Era stato ricoverato nel 1997, a 14 anni, in un centro di rieducazione per minori in seguito a diversi reati; nel 2006, un tribunale di Sibiu lo aveva condannato a 3 anni di reclusione per furto; graziato nello stesso anno, poco tempo dopo era partito per l'Italia. Questo soggetto viveva in Italia, non era tenuto a comunicare e a segnalare alle autorità italiane la sua permanenza. Le autorità di pubblica sicurezza non avevano alcuna possibilità di controllo, in quanto non esisteva ai propri atti il censimento di questo soggetto con tale fedina penale. n. 181 del 2007 viene annunciato con grande propaganda politica, sull'onda dell'emotività del Paese ed è finalizzato a porre lo Stato in condizioni di controllare meglio episodi ed atti di delinquenza come quelli compiuti da Mailat. Si scopre un grande deserto giuridico all'interno del quale dover intervenire, seppur nel rispetto delle direttive comunitarie, perché si tratta di disciplinare la permanenza di cittadini comunitari e non extracomunitari. La vicenda assume un tenore particolare perché ci si rende poi conto che da parte di cittadini comunitari scene o episodi simili a quello di Tor di Quinto si erano verificati il 17 agosto a Roma, vicino all'ippodromo di Tor di Valle dove un uomo di 60 anni era stato aggredito e colpito alla testa da alcuni rumeni; il 21 agosto a Roma tre rumeni avevano aggredito il regista Giuseppe Tornatore. Il problema esiste ed esplode nell'omicidio di Tor di Quinto. Ebbene, questo decreto, riconosciuto da tutti, è incapiente, inadatto a consentire al nostro Paese, alle nostre forze dell'ordine ed al nostro sistema di censire attentamente la platea dei cittadini comunitari, che vengono qui non tanto per turismo quanto per risiedere e, quindi, lavorare,

Come opposizione abbiamo svolto un ruolo estremamente responsabile; abbiamo votato i presupposti; stiamo facendo il meglio per migliorare il testo. Ci saremmo aspettati e ci attendiamo che su questi argomenti, che attengono alla salute e sicurezza dei cittadini, non vi potessero essere schieramenti da un lato e dall'altro, come temo si stia consumando in queste ore al Senato. Questo è il dramma del nostro Paese che sulla sicurezza, la maggioranza ed il Governo si stanno blindando per salvare se stessi, mettendo a repentaglio l'approvazione di un testo che, se migliore di quello attuale, sarà più efficace, migliore migliore per la tutela e la sicurezza dei nostri concittadini. Questo è il dato che pongo all'Assemblea. Dobbiamo dividerci sulla sicurezza?

che viene in Italia e che supera i tre mesi di permanenza, che si presuppongono permanenza per motivi turistici, di passaggio e non lavorativi, non destinati e finalizzati a radicare la propria residenza del nostro territorio, pone l'onere di pone l'onere di iscriversi nel registro anagrafico per motivi di sicurezza e di ordine pubblico perché iscrivendosi consente al nostro Paese di conoscere quella anamnesi del famoso Mailat, per esempio. Se il nostro Paese, il nostro Stato, le nostre forze di polizia avessero con questa norma conosciuto la storia di Mailat, probabilmente l'omicidio di Tor di Quinto non sarebbe avvenuto. Questo è il dato. Chiediamo questo; non altro, non chiediamo norme espulsive, sanzioni o condanne a morte. Chiediamo un sistema di censimento di chi entra in Italia. Vogliamo sapere chi è, cosa fa e la sua storia. Tutto qua! Il Governo pone un'altra norma, signor Presidente, che dice che questi soggetti, una volta superati tre mesi, possono - non debbono - comunicare alla questura la loro residenza e permanenza in Italia. C'è una bella differenza: o inseriamo una norma precettiva, un onere, un patto di lealtà tra l'altro tra il comunitario che decide di risiedere in un Paese che non è il proprio e quel Paese; un patto di lealtà, di conoscenza reciproca.

Allora vogliamo assumerci le responsabilità di questo testo e fare in modo che maggioranza e opposizione lavorino assieme per la sicurezza dei cittadini italiani o dividerci anche su questo tema, colleghi della maggioranza, del Governo, colleghi che intendono astenersi su questo voto? Io dico di no; sarebbe un errore. Vi è un Governo e una maggioranza in difficoltà, ne prendiamo atto, ma noi con il nostro atteggiamento, signor Presidente, collaborando in Commissione, abbiamo già detto, a voi ed al Paese, che non intendiamo strumentalizzare la sicurezza dei cittadini e questo decreto per la durata e la vita di un Governo ormai in agonia. Abbiamo detto che questo non c'entra, che non può costituire motivo di dibattito e di scontro politico; non strumentalizzeremo mai la tenuta del Governo a scapito della bontà di questo decreto e del suo eventuale

che gli italiani vogliono invece migliorato, perché ci tengono alla loro incolumità, e noi legislatori, noi eletti dai cittadini, abbiamo il sacrosanto dovere di assicurare loro migliore sicurezza e migliore tutela.

Signor Presidente, non oltrepasserò i cinque minuti. Ho ascoltato con interesse, come sempre, le osservazioni del presidente Schifani e vorrei dire che alcune cose sicuramente ci accomunano. Tanto ci accomuna la preoccupazione per il sentimento di insicurezza diffuso tra gli italiani, che rischia di generare sfiducia anche nelle istituzioni repubblicane, che noi siamo stati tra coloro che hanno sostenuto il Governo nell'adozione di una misura del tutto straordinaria, appunto dalla straordinaria necessità ed urgenza, come quella del decreto-legge che interviene in tale materia delicatissima della libertà della persone. Quindi, siamo d'accordo, è un problema serissimo con il quale la politica si deve confrontare anche con strumenti straordinari. Dopodiché, in questo momento ci occupiamo di un aspetto rilevante, ma minore. Si tratta, in sostanza, della possibilità di allontanare un cittadino comunitario che risiede in Italia per per più di tre mesi e che non abbia i mezzi necessari per il sostentamento e in qualche modo venga considerato di turbamento per la sicurezza del Paese. Vorrei ricordare che ciò è reso possibile nella disciplina dell'Unione Europea Europea per iniziativa impropria degli italiani. Come sappiamo, la storia della direttiva di cui ci occupiamo è legata al fatto che alcuni italiani, approfittando del regime particolarmente favorevole della Gran Bretagna sul terreno assistenziale, recavano in quel Paese e dopo i tre mesi si fermavano lì e usufruivano, in modo un po' improprio, dei benefici sociali che quel Paese consente alle persone che non hanno occupazione. A seguito di ciò nasce questa direttiva,

alla disciplina nazionale di prevedere che un cittadino comunitario che varchi la frontiera di un Paese debba in qualche modo registrarsi, che, anche per motivi di pubblica sicurezza possa essere imposto a questo cittadino comunitario,

Una norma così formulata è in esplicita violazione della direttiva. Oggi il collega Villone, secondo me molto chiaramente, ha spiegato che quella direttiva, essendo di immediata applicazione, costringerebbe il giudice italiano, chiamato a giudicare di un provvedimento di allontanamento, a disapplicare la norma interna in violazione della direttiva. Quindi, se votassimo oggi questo testo ci troveremmo nella situazione in cui il giudice non potrebbe poi applicare la relativa

Quale sia il contenuto di questa proposta lo ha illustrato il Governo e ricordato pochi minuti fa il presidente Schifani: il cittadino dell'Unione può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale e, se non lo fa, si presume che sia presente da più di tre mesi. Che cosa accade - lo chiedo al Governo - se il cittadino comunitario,

La situazione - vorrei dirlo al senatore D'Amico, il cui intervento ho seguito con attenzione - è diversa da quella del cittadino comunitario

la norma che prevede l'allontanamento, in questa ipotesi, parla di "cessazione delle condizioni" che determinano il diritto d'ingresso; ciò significa che il diritto di ingresso è già maturato, perché le condizioni si erano

avvocati civilisti - a me stesso: «Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie». Quindi, la direttiva permette di fissare il principio e prevede anche la possibilità di una sanzione: è esattamente quello che prevede il nostro emendamento. Rispetto a tale emendamento, vorrei dire

Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, su questo punto la discussione è stata assai lunga, in una Commissione che non ha potuto completare i propri ho cercato, in quella sede, di dire più volte che esiste una gerarchia delle fonti da cui non possiamo prescindere e che non possiamo inventarci una norma, anche con artifizi come quello di introdurre un riferimento alle misure di pubblica sicurezza, per violare direttamente e sostanzialmente una direttiva europea. Voglio leggere ai colleghi - perché a questo punto più di ogni argomentazione vale il testo - quello che dice il punto 11 dei *considerata* della direttiva europea di cui stiamo discutendo. Esso recita: «Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative». Noi non possiamo far dipendere dalle formalità amministrative, come l'iscrizione nel registro anagrafico, che comunque non ha nessuna funzione di pubblica sicurezza, il diritto a soggiornare nel nostro Paese ed è per quello che il Governo opportunamente ed alla luce proprio di quell'articolo 5, comma 5 della direttiva, invocato dal senatore Mantovano, ha introdotto il diritto a dichiarare la propria presenza da cui far discendere un'inversione dell'onere della prova. Credo, quindi, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, che al di là di ogni argomentazione retorica valgano i testi, da questi testi non possiamo prescindere e credo che a superare questo valga l'impegno del Ministro dell'interno a cercare di modificare la direttiva; ma credo che in nessun modo e in nessun caso possiamo nemmeno immaginare di poter cambiare la direttiva europea con delle leggi interne del nostro Paese. Per questo, signor Presidente, chiedo all'Aula di votare contro questo emendamento e di votare a favore di quello del Governo. *(Applausi

- «o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell'attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema d'iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell'interessato», si deve fare l'iscrizione anagrafica. Credo che questo possa

Vorrei dire che l'obbligo d'iscrizione anagrafica è già previsto nel decreto legislativo n. 30 del 2007. In particolare, è previsto, in termini chiari, all'articolo 9, comma 2, il quale dice testualmente che «l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso».

dopo i tre mesi - che è quella che autorizza il soggiorno dopo i tre mesi - si ritiene che esso stia nel territorio nazionale da più di tre mesi, salvo diversa prova contraria a suo carico. Assolutamente identica è la disposizione contenuta nell'emendamento 1.300 del Governo, il non ha dichiarato la sua presenza si ritiene che sia presente da più tre mesi, salvo prova contraria. Allora non comprendo davvero perché voi immaginate una norma di chiusura, che prevede la dichiarazione di presenza all'interno dei tre mesi, quando il soggiorno è completamente libero - e non la immaginate con riferimento al soggiorno dopo i tre mesi, quando il diritto non è più assoluto, ma è condizionato all'esistenza di determinati requisiti.

verrebbe sostanzialmente considerato come presente da più di tre mesi anche se vuole tornare a casa sua avendo finito il periodo di vacanza, mentre chi intende soggiornare oltre i tre mesi nel territorio nazionale soggetto ad un'analoga norma di chiusura. Vi renderete conto che questo è assolutamente irragionevole, alla luce della diversità del diritto di soggiorno pieno entro i tre mesi e del diritto di soggiorno condizionato, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva dopo i tre mesi. A me non pare che votare questa norma significhi portare acqua al mulino del centro-destra, piuttosto che fare uno sgarbo alla sinistra radicale; a me sembra che votare questo comma

dare alla dichiarazione di presenza di cui all'emendamento 1.300 del Governo.

e quindi il fatto che si possa ritenere che un cittadino comunitario stia nel nostro Paese da oltre tre mesi, quando c'è l'obbligo di dichiarare la propria residenza anagrafica. L'obbligo della propria residenza anagrafica scatta dopo i tre mesi. norma davvero singolare e totalmente priva di senso, perché dire che si inverte l'onere della prova e che quindi si presume che questo soggetto sia stato in Italia tre mesi, quando ormai tre mesi sono passati, credo sia un assoluto Ferma restando la considerazione sul fatto che questa norma non ha in sé alcun significato se non quello di complicare l'attività di accertamento sulla presenza degli stranieri nel nostro Paese, vorrei aggiungere, signor Presidente, che la norma che ha presentato il Governo con l'emendamento 1.300 (che invece pone l'inversione dell'onere della prova alla dichiarazione di presenza, cioè appena il cittadino straniero è entrato in Italia) è invece, quella sì, una norma che produce effetti giuridici,

perché fa presumere ciò che in realtà è già accaduto; dal punto di vista giuridico è largamente peggiorativa e inutile, e comunque largamente superata dalla norma

L'ho detto (lo ricordo bene) spiegando anche le ragioni: si chiede ciò che è già scritto nella legge, vale a dire che le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano con riferimento al documento d'identità si applichino anche al comunitario; la disciplina sui rilevi dattiloscopici cita espressamente gli italiani e quindi si applica anche al comunitario.

per gli extracomunitari che chiedono il permesso di soggiorno è previsto il rilascio dei rilievi fotodattiloscopici, per il cittadino italiano che chiede un documento di identità è previsto il rilascio dei rilievi fotodattiloscopici, per cui - afferma il Sottosegretario - per trasposizione delle norme per il cittadino italiano, ciò dovrebbe essere automaticamente previsto anche per il cittadino comunitario: perché allora non dirlo in chiaro? Capisco che c'è l'abitudine del Governo come dimostra l'emendamento 1.305 - di andare per sottintesi, però queste cose vogliamo che siano scritte non in un ordine del giorno ma in una legge dello Stato e nel modo più chiaro possibile

è evidente che, nel momento in cui si chiederà la carta di identità elettronica, non potrà che essere usata la stessa procedura per gli italiani e per i comunitari. È parimenti di tutta evidenza che, se si insiste per la votazione,

annuncia il voto favorevole (nel caso specifico su un certo emendamento) e poi vota in modo difforme rispetto all'annuncio che ha fatto, perchè questo è ciò che è stato fatto, un istante fa, da parte del senatore Sinisi.

nella disposizione: per rimanere oltre i tre mesi bisogna avere o un lavoro, o risorse lecite, o motivi di studio, o quant'altro è previsto dalla direttiva. Oltre i tre mesi, c'è inoltre l'obbligo di iscriversi all'anagrafe. Io ho messo insieme queste tre cose per individuare il comunitario buono che entra sul nostro territorio, segnala la propria presenza, si cerca un lavoro e, dopo i tre mesi, si dichiara all'anagrafe; dovessero venir meno questi requisiti, gli si segnala che entro un lasso di tempo deve abbandonare il territorio nazionale. Questa è l'ipotesi A: comunitario buono. Il comunitario cattivo,

dopo i tre mesi, non si iscrive neppure all'anagrafe. Credo che a questo punto vengano meno le riserve del collega Sinisi, secondo per mancata attuazione di fatti amministrativi non si può prevedere l'allontanamento. Io dico che una persona, se è entrata senza dichiararsi, non ha cercato un lavoro e non ha le risorse e se non si è iscritta all'anagrafe, si trova in una situazione di assoluta clandestinità (perché l'ha scelto lei);

permetta di distinguere i buoni dai cattivi e di liberarci dai cattivi, oggi ne abbiamo la possibilità, senza infrangere nessuna direttiva. Un auspicio: se è

però sia chiaro che è inutile stabilire che uno può dichiararsi, se poi non accade assolutamente niente. Purtroppo, tutto quello che abbiamo letto sulla cronaca nera dei giornali sarebbe comunque accaduto con il solo emendamento del Governo. (testo 3), perché segue questa strada. Chi decide di astenersi, quindi di estrarsi dalla tenzone, faccia il piacere di astenersi anche sull'emendamento

non so se ho sbagliato. In quel momento cercai di evitare che nei confronti di quel collega potesse essere irrogata una sanzione, perché era già stato richiamato all'ordine due volte.

sulla base non di quello che ho imposto io, ma che egli stesso aveva detto. Tant'è vero, senatore Schifani, che basta guardare gli atti del Senato (che mi sono riletto accuratamente)

argomenti abbastanza stravaganti, il dato fondamentale è molto semplice. Un senatore dell'opposizione ha dichiarato che avrebbe votato in un modo, ma poi ha votato in un altro. L'intervento della Presidenza è stato a dir poco autoritario,

assolutamente plausibile. Così non si può fare, signor Presidente, né vale - mi perdoni - il suo richiamo che siamo in ritardo. Non si possono cambiare le regole *ad libitum* perché si è in ritardo. Si rispettano le regole, che tra l'altro non si sa più quali siano

perché, come lei sa, al Senato come alla Camera, i precedenti hanno notevole importanza. Pertanto, mi ero procurato i precedenti della scorsa legislatura e volevo chiedere una testimonianza al presidente Pera; siccome, però, non lo vedo presente in Aula, non mi sembra opportuno intervenire.

non vorrei farmi qualche nemico, ma in politica capita - e desidero farlo con un esempio. Io faccio una dichiarazione a nome del mio Gruppo,

In politica - come dovrebbe essere - il parlamentare è libero di esprimere il suo voto come ritiene

al limite anche con un provvedimento, non so nemmeno di che tipo, ma nessuno può obbligare un senatore a votare come vuole il Presidente;

il mio disagio, e quindi il mio dissenso. Infatti, una votazione di elementi così smembrati, a mio avviso, fa venir meno

Capirà, Presidente, che è un po' strumentale, ma anche il sottoscritto dichiara di votare in dissenso rispetto al Gruppo. La mia è una provocazione ancora più forte, perché le

riguardanti il tema della sicurezza che trattiamo, evidenziando il fatto che lo Stato oggi non sa garantire la domanda di sicurezza che viene dal Paese.

Quali sono le loro azioni? Ognuno si difende come può: mette le barre alle finestre, installa i sistemi di video-sorveglianza, si attrezza in modo da autogarantirsi quella sicurezza che lo Stato non gli garantisce. In Aula abbiamo presentato emendamenti che andavano in questa direzione, sistematicamente bocciati dal relatore e dal Governo. È possibile che lo stesso Governo, la stessa maggioranza blocchino dei provvedimenti al Senato e li approvino poche settimane dopo alla Camera? È inconcepibile ed inaccettabile. Questa è la motivazione della nostra protesta e del dissenso strumentale, che servirà a trovare una regola, finalmente unitaria, non *bipartisan* e non unilaterale, sulle dichiarazioni e sui voti conseguenti della libera determinazione, che deve sempre rimanere in capo al singolo senatore.

non mi soddisfa completamente l'emendamento del collega Calderoli, nonché vice presidente del Senato (se capisco la *ratio* della sua

nell'emendamento sia la cosa più opportuna da fare; onestamente, faccio fatica a capire anche la posizione del Governo e dei colleghi di maggioranza, proponenti il provvedimento in esame, dal momento che vi è stata nelle ultime settimane un po' di confusione da parte della maggioranza e del Governo stessi. Intanto, da abitante della provincia di Varese, non posso non sottolineare che, con rispetto per tutti i cittadini e soprattutto con il massimo rispetto per le vittime, se non fosse successo un così grave fatto di sangue nella città di Roma non si sarebbe addivenuti assolutamente a nulla. nulla. Potremmo ricordare che nei mesi precedenti - il 10 ottobre, il 21 agosto, il 22 settembre e il 6 marzo di quest'anno - ci sono stati delitti altrettanto violenti, cruenti, efferati, che hanno comportato una quantità notevole di vittime nelle Regioni padane, di fronte ai quali da parte dello Stato non vi è stata la minima reazione, se non quella di mandare avvisi di garanzia

quanto ha fatto adesso la Lega, perché credo abbia fatto bene a denunciare una prepotenza che si sta verificando in quest'Aula. Per quel che mi riguarda, dichiaro il voto in dissenso dal senatore Sinisi, in attesa che si decida a fare quanto dice.

lei ha concesso la parola a quei colleghi sulla base della dichiarazione di voto in dissenso dal loro Gruppo. Le faccio notare che questa è una norma di garanzia per i lavori dell'Aula ed è esattamente una norma antiostruzionistica. È cioè finalizzata a garantire il corretto funzionamento del nostro Senato, perché è una norma violando la quale le discussioni non potrebbero mai avere fine.

Ora, giustamente, il senatore Castelli aveva espresso la sua opinione a nome del suo Gruppo. Dopodiché, sono intervenuti - perché il collega Castelli e i colleghi della Lega Nord conoscono perfettamente il Regolamento

- il Gruppo della Lega Nord ha violato una norma del nostro Regolamento. Glielo volevo far notare, perché lei non lo aveva notato.

che va affrontato in maniera seria e sul quale bisogna trovare una posizione definitiva. Per questo ritengo necessario un momento di riflessione in Giunta per il Regolamento.

Cercherò, per parte mia, di essere lucido, e mi auguro che voi non siate sordi. L'emendamento 1.300 del Governo - vi piaccia o no - è contrario alla direttiva europea

«Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale». Quindi, lo Stato membro può obbligare l'interessato ad effettuare la dichiarazione di presenza, nell'emendamento 1.300 non vi è alcuna previsione d'obbligo, ma si ipotizza una facoltà. In secondo luogo,

non vi è alcuna indicazione di un termine ragionevole e non discriminatorio entro cui effettuare tale dichiarazione, con la conseguenza che, se non viene effettuata entro giorni uno dall'ingresso nel territorio nazionale,

In altri termini, non siamo sfavorevoli a che voi, oltre a richiedere l'iscrizione anagrafica - già prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007 - imponiate anche la dichiarazione di presenza,

avete paura d'inserire, sia nell'obbligo di iscrizione, sia nella dichiarazione di presenza, il termine «pubblica sicurezza». la dichiarazione di presenza, così come la richiesta anagrafica, senza il riferimento ai motivi di pubblica sicurezza non serve assolutamente a nulla, perché quando vi imbatterete nel Mailat di turno, che non ha ottemperato all'obbligo di iscrizione o non ha ottemperato alla dichiarazione di presenza, non sarete assolutamente in grado di provvedere al suo allontanamento.

si inserisce, così come è stato congegnato, nel testo del decreto di recepimento della direttiva il quale già contiene, come è stata ricordato anche dal senatore Palma, all'articolo 9, l'obbligo di dichiararsi, ma a differenza della terminologia estremamente generica della prima parte dell'emendamento 1.300 del Governo, fissa una conseguenza in caso di omessa dichiarazione. Credo che questo emendamento sia molto più in linea con il decreto di recepimento e quindi con la direttiva rispetto all'emendamento del Governo e approfitto, signor Presidente, proprio perché è un dato esclusivamente tecnico, per chiedere ai colleghi del centro-sinistra, anche in questa votazione, di non farsi guidare da pregiudiziali ideologiche. Questo decreto si sta formando con

ecco a cosa conduce la pregiudiziale ideologica che sta animando il centro-sinistra nell'esame di questo provvedimento. Stiamo tentando di migliorare l'emendamento del Governo; mi auguro che questo tentativo di miglioramento abbia un esito diverso rispetto agli emendamenti precedenti.

Presidente, ma quello che le dirò è di estremo interesse politico, anche perché mi rivolgo a lei, signor Presidente, e spero che presti attenzione anche la sottosegretario Lucidi.

ha espresso disappunto per il respingimento di alcuni extracomunitari iracheni e afghani verso la Grecia dai porti dell'Adriatico.

la prassi di respingere dai porti adriatici i rifugiati iracheni e di altre nazionalità verso la Grecia. Ora, domando a lei, signor Presidente, e alla sottosegretaria Lucidi per quale motivo le autorità italiane hanno dato disposizione di bloccare indiscriminatamente - così com'è avvenuto - tutti i respingimenti ai valichi di frontiera di qualsiasi sedicente rifugiato politico, soprassedendo ad ogni tipo di puntuale controllo sulla sua provenienza o sull'effettivo *status* di rifugiato. Questo vorremmo saperlo, perché se il Governo comincia a dare disposizioni di una semplice richiesta da parte di un'associazione qualsiasi di bloccare qualsiasi respingimento (anche quello, ad esempio, dei fantasmi che vogliono venire a inondare le nostre lande), allora siamo veramente allo sbando.

stiamo dimostrando a cosa si può arrivare se le regole non vengono rigorosamente rispettate ogni volta e non in funzione della convenienza dell'Aula. Questo è il dato che noi ci premuriamo di dimostrare.

il diritto del senatore fino a quando non ha espresso il voto non è coartabile. Qualcuno di voi ha richiamato un episodio, che è stato chiarito dal senatore Angius, al quale è stata data una connotazione diversa - così é stato ritenuto - che impone un chiarimento. Il chiarimento chiarimento si può avere soltanto nell'ambito della Giunta per il Regolamento trattandosi di un argomento di rilievo costituzionale e non soltanto regolamentare, che non può essere affrontato nell'ambito di una polemica di carattere prevalentemente politico. Questa è la posizione che ho espresso e che assolutamente, in coscienza, non intendo cambiare; per questo ora dico che non forziamo niente.

Questa è la regola generale che abbiamo applicato e discusso molte volte; non entra in gioco oggi pomeriggio.

Faccio riferimento proprio alla questione con la quale lei intende impedire la manifestazione del dissenso. Prima il presidente Matteoli - cercherò di non aggettivare il mio intervento argomentazioni ha sostenuto che il senatore, fino al momento del voto, ha anche il diritto di cambiare opinione, perché il dibattito può farla mutare. Presidente, lei qui dispone verso i dissenzienti, ma anche se capiamo quanta strumentalità ci possa essere in un atteggiamento (ma si tratta di una scelta politica che lei non può mettere in discussione, perché lei presiede il Senato e non capeggia l'opposizione), lei deve consentire a quei colleghi di esprimere la loro protesta. Anche perché lei, in questa giornata, in questa seduta, ha omesso - questo è il difetto del ragionamento del presidente Angius - di censurare l'atteggiamento del collega Sinisi. Non interveniva in dissenso, il senatore Sinisi, ma è intervenuto in dissenso dopo l'intimidazione del presidente Salvi riferita al mancato parere del Governo. Questo è quanto è successo in Aula. Lei non ha garantito il diritto del senatore Sinisi a poter votare, come aveva annunciato, a nome del Gruppo più importante di quest'Aula. Signor Presidente, il senso del mio intervento sul Regolamento è il seguente. Ella ha annunciato che convocherà la Giunta per il Regolamento. Giustissima decisione. Signor Presidente, nessuno può già stabilire quale sarà la decisione della Giunta per il Regolamento, quindi delle due l'una: o lei convoca immediatamente la Giunta per il Regolamento per dirimere la questione o consente di continuare nell'atteggiamento fino a che non sia contraddetto da una deliberazione della Giunta.

è una domanda alla quale non chiedo risposta: qual è l'articolo del Regolamento che consente, come ha fatto il presidente Angius quando presiedeva l'Assemblea, di togliere la scheda ad un senatore presente in Aula? Quando il senatore Angius mi dirà qual è l'articolo che lo permette... Concluda, per favore.

signor Presidente, c'è una questione sulla quale dobbiamo fare chiarezza. Il voto in dissenso è stato disciplinato dal Regolamento e poi dalla prassi perché veniva utilizzato come forma ostruzionistica per allungare i tempi del dibattito, non c'era altro motivo.

va benissimo la prima decisione, ma dissentiamo che si consenta di utilizzare tempi ulteriori rispetto a quelli che la Conferenza dei Capigruppo, all'unanimità,

d'ufficio, ma vorrei significare alla Presidenza - e l'avevo manifestato nel mio precedente intervento - il malessere di un'opposizione che riscontra nella Presidenza una gestione secondo la quale, a seconda chi compie un determinato gesto, si è o non si è nelle regole. Questo è il tema che la Presidenza avrebbe dovuto evitare. Quello che ci ha preoccupato di più non è soltanto questa anomalia, ma la velocità - non mi permetto di dire leggerezza, signor Presidente - con cui la Presidenza ha cercato di andare avanti su quell'episodio. Sono certo che il Presidente fosse al corrente del passato trascorso della presidenza Angius;

ricorso ad un ostruzionismo al quale non ricorre spesso. Devo dire che in questa occasione, così come in occasione della finanziaria e di altri testi importanti, non mi pare che quest'Aula sia stata caratterizzata da atteggiamenti ostruzionistici. Quindi, nel confermare il nostro impegno, non posso che ribadire, signor Presidente, la preoccupazione e il malessere di questa opposizione. Ritengo e mi auguro di poter rappresentare il malessere dell'intera opposizione, non soltanto della Lega, che lo manifesta in altro modo. Ma il malessere c'è, signor Presidente. Lei non può continuare a gestire l'Aula decidendo in senso unilaterale, per poi scaricare le decisioni assunte *ex post* - come diceva la collega Alberti Casellati - ad una Giunta che quasi sempre decide con il voto determinante della sua persona, così come è sempre Allora, delle due l'una. Dobbiamo porci attentamente questo tema. La Lega lo sta ponendo in questo modo. Io mi auguro, e lo dico con grande responsabilità, che si eviti al Gruppo di Forza Italia di dover seguire ed imitare in futuro il percorso della Lega;

la parola data e il rispetto dei patti. Il collega Boccia ha dichiarato che, in qualche modo, le dichiarazioni del senatore Schifani avrebbero dovuto coinvolgere tutta l'opposizione. Capisco che il collega Boccia - anche legittimamente, dal suo punto di vista - è in questo momento permeato da una *cupio* bipartitica, per cui c'è un grande partito a sinistra e un grande partito a destra, però, al momento, le cose non stanno così; per il Gruppo della Lega

soprattutto in questa legislatura l'interpretazione, che pesa su come comportarsi in relazione al voto dei singoli senatori, è molto incidente su quello che può essere il risultato politico. Noi abbiamo assistito ad una interpretazione da parte della Presidenza che non ci aveva convinto. C'è stato anche un dibattito molto approfondito sul tema.

annunci e delle dichiarazioni di voto. L'articolo 110, invece, parla degli interventi nel corso della votazione e fa riferimento ai casi specifici nei quali la Presidenza può intervenire o durante i quali si può mettere in discussione il voto. D'altronde, non potrebbe essere diversamente, perché il voto del singolo senatore è protetto da una norma costituzionale e nessun Regolamento può incidere o pesare nel momento dell'espressione del voto.

D'altronde questo è il sale della democrazia. La democrazia si basa sulla possibilità concessa a ciascuno di cambiare opinione e soprattutto sul fatto che quando si vota si presuppone che il voto non sia l'affermazione

Capisco che possa esservi un dissenso per quanto riguarda le conseguenze regolamentari di un comportamento diverso dall'annuncio fatto,

nel caso in cui c'è un comportamento difforme da quanto dichiarato, fermo restando che il voto rimane nella libera e assoluta disponibilità del senatore.

non garantisce l'esistenza della libera manifestazione di volontà dei senatori non è più uno strumento di democrazia

che su questo problema non sono in discussione i princìpi, sui quali siamo tutti d'accordo, ma la necessità di approfondire la questione in relazione alle fattispecie che si possono presentare, ribadisco, al di là delle parole che ho sentito, che la volontà della Presidenza di prendere decisioni legate alle posizioni politiche o personali che si esprimono è al di fuori da ogni mia preoccupazione. Quindi, su questo piano, vedo solo quella via d'uscita. Vi pregherei di riprendere le votazioni, con ordine, perché siamo fortemente in ritardo; questo è un argomento per il quale abbiamo scadenze molto stringenti, come atto di responsabilità del Senato.

posto: vediamo se riusciamo a far ripartire i nostri lavori.

nell'emendamento che propone il Governo s'immagina una semplice facoltà comunitario di dichiarare la propria presenza. Signor Presidente, se io fossi un comunitario e lei fosse lo Stato italiano, tradotto in termini molto concreti, quasi caserecci, ciò

bussare. Questo emendamento, allora, punta a trasformare una facoltà in un obbligo: se desidero entrare a casa sua, busso; lei chiede che mi qualifichi, dopodiché, se vi sono le condizioni per entrare, entro. Non è vietato dalla direttiva comunitaria, perché questa si occupa di un diritto di soggiorno già maturato: qui non vi sono ancora le condizioni che hanno fatto maturare il diritto di soggiorno e neanche quello di ingresso. poi è necessario che vi sia l'obbligo? Immaginiamo - cosa tutt'altro che contraria alla realtà - che un soggetto comunitario abbia precedenti, in Italia o nel proprio Paese: la dichiarazione consente all'autorità di pubblica sicurezza di verificare tali precedenti e, se esistono motivi imperativi di sicurezza (e ciò spiega il collegamento dell'obbligo al richiamo a tali motivi), di decidere chi non ha titolo per stare qui. Vorrei capire perché un emendamento di così elementare buon senso debba essere bocciato. L'emendamento 1.300/2 dovrebbe essere votato unitamente all'emendamento 1.300/4 della senatrice Thaler

sostituire il termine "può", facoltà dell'interessato, con il termine "deve", obbligo dell'interessato.

dichiara: «Non ricordo precedenti nel mondo politico, quantomeno occidentale, in cui lo *speaker* di un ramo del Parlamento entri a piedi uniti sulla situazione politica attuale colpendo direttamente il Presidente del Consiglio in carica. Purtroppo anche questo è il segno di un ricorrente e diffuso affievolimento del senso dello Stato». Lo afferma

dichiarazione non è un esponente dell'opposizione e nemmeno un collega della maggioranza, ma è addirittura un uomo che fa parte del Governo. Credo che una

richiamandosi al buon senso e credo che in quest'Aula nessuno possa ignorare quanto ha detto. Come senatore vorrei avere una risposta dal Governo. Il sottosegretario Lucidi in questo dibattito

dite che si può fare proprio secondo la direttiva comunitaria. Noi vi chiediamo di dire che si deve fare secondo la direttiva comunitaria. Vorrei avere una spiegazione sull'incaponimento del Governo nel rifiutare una norma di buon senso che garantisce finalmente e per sempre i cittadini italiani.

per dichiarare la presenza del cittadino comunitario nel nostro Paese sia ritenuta valida anche quella effettuata dai soggetti

non riesco a pensare come un ordine del giorno possa tradurre il termine «può» con «deve»: o l'ordine del giorno parla di altro, quindi è inammissibile,

però dichiara in modo esplicito: «deve dichiarare ad un ufficio di polizia» secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero. Pertanto, se il decreto del Ministero stabilisce

*(FI)*. Intendo dire questo e lo ripeto dall'inizio: non so se, come cofirmatario, posso interloquire. Fin d'ora le dico, però, Presidente, che se gli altri firmatari sono

Signor Presidente, avevo chiesto la parola sull'emendamento 1.300/4 (testo 2) intanto per poter leggere l'ordine del giorno perché non credo sia un fatto privato tra il Governo ed il presentatore dell'emendamento e quindi per poterci regolare di conseguenza; in secondo luogo, chiedo al Governo - mi sembra quasi offensivo nei confronti dell'Assemblea fare questa domanda ma non lo è nei confronti del Governo - se siamo arrivati al punto che giuridicamente la facoltà è assolutamente parificata all'obbligo.

È possibile che la facoltà sia parificata a un dovere? È possibile trasformare un emendamento - in cui si dice che non basta la mera facoltà, ma ci vuole l'obbligo - in un lunghissimo ordine del giorno assolutamente incomprensibile, che soprattutto non dà conto della finalità dell'emendamento, che non era quella di lasciare alla discrezionalità soggettiva ma di fissare un obbligo di lealtà nei confronti dello Stato? Le chiedo allora di leggere l'ordine del giorno e di valutare la sua ammissibilità sotto il profilo della assoluta diversità

un ordine del giorno che inserisce un principio irrazionale, assurdo ed inaccettabile! Capisco, colleghi, che avete problemi di tenuta, però, vivaddio, non offendiamo la regola della razionalità legislativa. A tutto c'è un limite!

andando al di là di ogni logica politica e giuridica, però a tutto c'è un limite, Presidente. Io chiedo, credo a buon diritto, di conoscere il testo di questo ordine del giorno per poterne discutere.

nuova finestra") Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1872 di conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, impegna il Governo a prevedere che tra le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno per dichiarare la presenza del cittadino comunitario nel nostro Paese sia ritenuta valida anche quella effettuata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 109 del regio

qual è la modalità di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza (e se il Governo ha la bontà di ascoltare, poi avrà la bontà doppia di rispondere). In secondo luogo, se vale la prima parte di questo atto di impegno, questa stabilisce semplicemente delle modalità di presentazione di una dichiarazione, cioè come deve essere fatto il modulo, davanti a chi deve essere presentato, se con timbri o senza timbri e così via, ma non scioglie assolutamente il quesito dal quale siamo partiti e cioè se è una facoltà o un obbligo. Quindi, signor Presidente, a mio avviso, non risolve il problema di sostituire l'emendamento presentato che, quindi, non può essere surrogato dal presente ordine del giorno.

Ausserhofer, non sarò colpito negativamente dal suo bellissimo richiamo legislativo, ma vorrei capire: i destinatari del regio decreto del 1931 erano cittadini comunitari?

da cui si desume che abbia accettato che il senatore Palma diventasse cofirmatario dell'emendamento. È di tutta evidenza che la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno richiede l'approvazione anche del senatore Palma.

seconda questione, sollevata anche dal senatore Storace, sta nel fatto che è del tutto evidente che la trasformazione in ordine del giorno è valida se rispecchia fedelmente - e direi quasi pedissequamente - lo spirito e la forma dell'emendamento. Se lei, signor Presidente, consente - come mi pare di aver capito da alcune sue espressioni,

ma è un ordine del giorno, quindi una cosa diversa, chi accetta l'invito alla trasformazione ha anche una sua discrezionalità nell'accettare la dizione. Questi sono i comportamenti che abbiamo sempre tenuto.

fare propria una volontà, che era quella di trasformare una facoltà in un obbligo; vorrei capire come un ordine del giorno possa essere in sintonia con questa strategia. Vorremmo, ripeto, conoscere

1.300/3, vorrei dire, per essere molto chiari, che il Governo ha dato parere favorevole all'ordine del giorno così come formulato dalla senatrice Thaler

che le dichiarazioni che devono essere fatte, sia pure da altra persona (gli albergatori), si ispirano alle ragioni di pubblica sicurezza che sono ricomprese

poiché il Governo aderisce all'ordine del giorno della senatrice Thaler Ausserhofer, che invero fa riferimento ad una dichiarazione di presenza per interposta persona, credo che analogamente non abbia nessun problema a riformulare il suo parere in ordine all'emendamento

che si trova nel Testo unico di pubblica sicurezza e che si ispira a ragioni di pubblica sicurezza; siccome il Governo si è pronunciato favorevolmente e forse addirittura, in qualche modo, ha stimolato, attraverso l'invito al ritiro, la formulazione dell'ordine del giorno, io non credo davvero che il Governo

«I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti». Questo è il riferimento che viene fatto.

che occupano gran parte delle nostre discussioni, ma poiché la Presidenza questa volta ha guardato da questa parte sono in grado ora di intervenire anche io. Penso che l'ordine del giorno, così come del resto è stato spiegato dal presidente Marini, offra una garanzia in più alle persone che soggiornano nel territorio nazionale e che sono stranieri appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione. Questa garanzia in più consiste nel fatto che vale come dichiarazione della propria presenza anche l'attestazione da parte di quei soggetti citati nell'articolo del testo unico. Vorrei per un momento solo respingere la tesi suggestiva, proposta qui dal collega Mantovano e poi ripresa anche con enfasi dal presidente Schifani, secondo la quale con con il subemendamento 1.300/3 si compie una scelta decisiva ed assai importante ai fini della determinazione di questa norma poiché con essa si passa dall'affermazione di una facoltà all'affermazione di un obbligo. Questo subemendamento, collega Mantovano, è in realtà di scarsissima rilevanza poiché l'emendamento 1.300, che il subemendamento vorrebbe correggere ed integrare, stabilisce un meccanismo che il subemendamento, comunque, non tocca e che è strutturato in due momenti: lo straniero soggiornante in Italia segnala la sua presenza con un esplicito riferimento ad una previsione di durata del soggiorno. Quali sono le conseguenze della segnalazione della propria presenza? Che per tre mesi egli potrà esercitare il diritto di soggiorno senza alcun problema, in modo del tutto libero e senza che si ponga la questione delle proprie fonti di sostentamento. Allo scadere del terzo mese si apre un regime diverso, nel quale l'autorità prefettizia può valutare che l'assenza di risorse e la nullatenenza di questo soggetto - unita ad altre valutazioni, poiché essa da sola non basta - fa venire meno le condizioni per l'esercizio del diritto di soggiorno. Qui davvero la pubblica sicurezza non c'entra nulla, poiché è evidente dalla direttiva europea, così com'è evidente dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che il problema centrale è far sì che la persona straniera che risiede in Italia non gravi sull'assistenza pubblica, non si trovi in una condizione di assenza di fonti di sostentamento; se, infatti, si trova in questa condizione il prefetto può disporre l'allontanamento, anche se

Il decreto-legge stabilisce anche un effetto della mancata ottemperanza all'allontanamento, che è rappresentato dall'obbligo, dal dovere di vidimazione di un documento, consegnato allo straniero che deve essere allontanato, presso il consolato italiano del suo Paese di origine. Questo è l'unico obbligo che si può stabilire, poiché sulla base della direttiva europea non si potrà stabilire un divieto di reingresso. Il decreto-legge, in questo caso è chiaro. La segnalazione della propria presenza è indicata con il "può" poiché si tratta di un onere finalizzato all'esercizio del diritto di soggiorno. E che significa "può"? Che se non lo fa, se non segnala la propria presenza, nel momento in cui si effettua un controllo si ritiene, fino a prova contraria, che egli sia in Italia da più di tre mesi: ecco come funziona il meccanismo dell'onere. allora di accantonare concetti di teoria generale del diritto civile, come "facoltà" od "obbligo", perché in questo caso non si tratta né di una facoltà né di un obbligo, ma ci troviamo di fronte

Quindi, tutto il resto, cari colleghi, sono divagazioni sul tema, divagazioni incongrue che si scontrano con lo spirito e anche con la lettera della direttiva europea e del decreto legislativo che da essa è nato.

emendamento in ordine del giorno non spetta né al Governo né al presentatore, ma alla Presidenza, e devo ammirare la sincerità dando successivamente lettura del riferimento normativo perché il suo giudizio è stato espresso prima ancora di conoscere il contenuto. Ora abbiamo avuto conoscenza da lei del contenuto. Voglio rileggere quello che c'è scritto nel subemendamento originale, che prevede di sostituire le parole: «può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare» con le seguenti: «deve dichiarare ad un ufficio di polizia».

prima è una questione per regolare gli ingressi e dar conto dei presenti, l'altro è per venire incontro agli albergatori. Mi sembra veramente troppo.

una facoltà ed un potere del genere. Su una polemica particolaristica stiamo mettendo in discussione un principio fondamentale del procedimento legislativo. Questa è la mia profonda convinzione.

Presidente, che c'è un diritto del presentatore dell'emendamento, ed è sicuramente vero. Non c'è però il diritto del presentatore dell'emendamento a

Signor Presidente, lei sa che ci applichiamo molto ad estraniarci da quello che avviene in Aula, perché è importantissimo il lavoro che svolgiamo, ma le agenzie di stampa ci consegnano senza enfasi un quadro che rende questo nostro discorso

E aggiunge (ed è la nota che vorrei sottolineare): a questo gioco non ci sto, qui al Senato sono mancati 400.000 voti, forse è irregolare la nostra stessa maggioranza. Sono parole che nemmeno l'opposizione ha mai usato per definire il Senato a cui il Ministro della giustizia, essendone membro, ricorda che la maggioranza qui non c'è perché elettoralmente sono mancati 400.000 voti. Nella deprecata Prima Repubblica, alla cui ragione sociale si richiama il mio partito, dopo l'intervista di Bertinotti il Governo si sarebbe dimesso, invece in questo caso fa rispondere ad un Sottosegretario importante che il presidente Bertinotti è in errore,

All'opposizione rimane la soddisfazione di sentir dire per la prima volta da un membro di quest'Aula, che è Ministro e *leader* importante della maggioranza, che questo Senato ha una maggioranza irregolare: la per oggi all'opposizione può bastare anche questo. perché la questione mi è sembrata - lo dico alla collega Thaler Ausserhofer - onestamente un po' il gioco delle tre carte e io non vorrei concorrere a trasformare l'Aula del Senato nel gioco delle tre carte, che è un illustre ed importante gioco che si svolge a Napoli. Non so se la collega Thaler Ausserhofer intende partecipare a questo gioco. Faccio una domanda alla collega. Non ho nessuna intenzione di percorrere le notevoli questioni regolamentari e costituzionali che sono state avanzate; sono tutte molto serie, non meritevoli di diventare il gioco delle tre carte. Ho avuto carte. Ho avuto il testo dei subemendamenti. Mentre vedo il nostro subemendamento (Schifani, Matteoli, D'Onofrio ed altri) scritto in stampatello, poi vedo scritto, non ho capito con la grafia di chi (vedo "Thaler"),

dicono di no. Allora vuol dire che è un documento falso. Ecco perché è il gioco delle tre carte. Vorrei capire la collega Thaler Ausserhofer cosa ha scritto come subemendamento. Quello che ho evidentemente è un falso, se la collega Thaler Ausserhofer dice che non ha detto questo; vuol dire che abbiamo un documento falso. Vorrei capire di cosa stiamo discutendo.

"può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare" con le seguenti: "deve dichiarare ad un ufficio di polizia"». Per carità! La collega Thaler Ausserhofer vedo che capisce anche l'italiano, ne sono molto lieto.

Infatti, il suo subemendamento, anziché dire, come io credevo, che «può» deve essere sostituito con «deve», dice che «può presentarsi» deve essere sostituito con «deve dichiarare». Per carità, capisco che non sono esattamente la stessa cosa. Nel gioco delle tre carte sarebbero considerate la stessa cosa; non so se la collega Thaler Ausserhofer il gioco delle tre carte lo conosce o no. Nell'ordine del giorno scritto

per dichiarare la presenza del cittadino comunitario nel nostro Paese sia ritenuta valida anche quella effettuata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773». La collega Thaler Ausserhofer sa cosa dice questo decreto,

Di una cosa sola sono certo:

molti colleghi avanzano argomentazioni pretestuose che non hanno a che fare con il merito della discussione), che abbiamo un subemendamento presentato

No. Immediatamente dopo dobbiamo discutere e votare un emendamento che è esattamente identico. Non capisco quindi di cosa stiamo discutendo. La senatrice Thaler ha ritirato il proprio subemendamento e ha proposto un ordine del giorno che il Governo ha accolto, adesso diamo soddisfazione al collega Nitto Palma e discutiamo l'emendamento

«All'emendamento 1.300, sostituire le parole "può presentarsi" con le seguenti "deve dichiarare per ragioni di pubblica sicurezza".

Signor Presidente, ovviamente seguo l'*iter* logico che lei ha esposto a proposito dal rapporto tra emendamento e ordine del giorno; pur non condividendolo, non lo discuto. Vorrei soltanto esporre, in sintesi, i punti essenziali dell'emendamento in discussione. In quell'ordine del giorno, si affronta il tema dell'obbligo dei gestori di alberghi, di campeggi, di proprietari di case che le affittano e così via. Non riesco allora a capire per quale ragione logica, nel momento in cui si pone e si richiama quest'obbligo in capo ai gestori, conseguentemente uno in capo a coloro che devono presentare quella dichiarazione ai gestori, che poi la trasmettono all'autorità di sicurezza.

necessariamente deve esservene uno del cittadino comunitario che consenta ai primi di adempiere al proprio. Per concludere, l'insieme Per concludere, l'insieme dell'ordine del giorno non soddisfa l'emendamento della senatrice Thaler Ausserhofer; da ciò la necessità di votare questo emendamento, perché, se il problema è apparentemente risolto, con riferimento ai cittadini comunitari che prendono una stanza d'albergo o una *roulotte* in un campeggio, non lo è con riferimento ai cittadini che entrano, ma non alloggiano in nessuna struttura per la quale il gestore sia obbligato a presentare la propria dichiarazione. Rispetto a tale posizione, poiché l'ordine del giorno Thaler Ausserhofer, sostitutivo del suo emendamento, non dà alcuna risposta, è obbligatorio, per coerenza con coloro che hanno condiviso l'ordine del giorno precedente, votare a favore del presente emendamento.

nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ciò significa che tali motivi vengono in considerazione per questa disciplina. Per le suddette ragioni voteremo a favore del subemendamento.

è stato trasformato in un ordine del giorno, vorrei che lei invitasse il presidente della Commissione bilancio, senatore Morando, a convocarla subito. trattandosi di alberghi, ostelli e campeggi dell'Alto Adige, non vorrei che sotto vi fosse qualche finanziamento per quelle zone. La prego di voler invitare la Commissione a verificare chevi sia la copertura finanziaria*.

comma 7 dell'articolo 95 parla della trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno. Lo faccio, colleghi, a garanzia di tutti, della maggioranza e dell'opposizione, che si alternano in un sistema - per fortuna - bipolare. Presidente, leggo il comma 7: «Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione» - perché naturalmente non si tratta altro che dell'emendamento stesso presentato nei termini e trasformato in ordine del giorno - «e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo che l'ordine del giorno in cui è stato trasformato un emendamento è sottoposto ai limiti previsti per gli emendamenti. Presidente, uno di quei limiti, sotto il profilo dell'ammissibilità, è la coerenza del suo testo con il testo principale in cui si va ad inserire. sostanza, non si può presentare un emendamento di carattere economico su un testo ordinamentale. Non si può presentare un emendamento che parla di sanità ad una legge della giustizia. Conosciamo tutti la logica della coerenza delle proposte emendative sul testo base. A questa stessa coerenza il comma 7 dell'articolo 95 richiama proprio l'ordine del giorno, in quanto deve essere compatibile e coerente con il testo nel quale si inserisce, ossia con l'emendamento del quale è trasformazione.

che è un *vulnus* per la nostra Aula. La proposta di ordine del giorno in questione non contiene affatto - dico affatto - alcun principio dell'emendamento della collega Thaler, il quale mirava a trasformare una facoltà in un precetto, in un obbligo. L'ordine del giorno dice tutt'altro. Allora, se lei vuole non solo innovare la prassi, ma anche non rispettare il Regolamento, dichiarando ammissibile la trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno che contiene un principio completamente diverso, compie una irregolarità. Dico anche che la collega Thaler - secondo il mio modesto parere - farebbe bene a ritirare l'emendamento e l'ordine del giorno anziché tenere l'Aula bloccata su una procedura irregolare, inammissibile, inaccettabile. *(Applausi verità. Non intendiamo minimamente abbassare la guardia allorquando vengono calpestate non soltanto le prassi, che sono anche fonti, ma le stesse norme regolamentari alle quali ci siamo attenuti in tutti questi anni, sia quando eravamo maggioranza che quando eravamo opposizione. Lei non troverà mai, Presidente, un precedente di un emendamento trasformato in ordine del giorno che va in direzione diametralmente diversa - non dico opposta - rispetto alla volontà emendativa. Allora, Presidente, insisto per conoscere attentamente la volontà indicata nell'ordine del giorno e la sua compatibilità con l'emendamento del quale sarebbe - dico sarebbe, perché mi rifiuto di accettare che sia stato dichiarato ammissibile - la trasformazione. finestra"). Prendo atto dell'opposizione fermissima e di tutto il resto. Se le modalità sono rispettose delle regole, il Presidente sa bene che poi può essere soggetto a fortissime contestazioni. Può capitare

dagli atti. Mi fermo qui perché la decisione è stata quella: lo fermiamo e andiamo avanti, però, qui non si tratta di materie diverse, ma di diverse modalità - almeno questo è il mio giudizio in detto momento - di rispondere alla stessa esigenza.

L'articolo 5, comma 5, di quella direttiva stabilisce che: «Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza»;

decorra già da tre mesi. Pertanto, se diamo una facoltà e non prevediamo un obbligo di fare tale dichiarazione, non aiutiamo il cittadino comunitario,

Vorrei conoscere il parere del Governo su questo emendamento terribile, che sconvolge il decreto e che stabilisce semplicemente un termine per il Ministro dell'interno per emanare un decreto ministeriale. PRESIDENTE. Il parere

prescrive l'obbligo di dichiarare la presenza deve, altresì, stabilire un tempo congruo e ragionevole. Se non viene prescritto alcun termine per fare la dichiarazione, evidentemente basterebbe un solo giorno

si vada a leggere l'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, dove si prevede l'allontanamento del cittadino dell'Unione, esattamente perché sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 7, che sono, per l'appunto, tutti requisiti economici.

avevo chiesto già da prima la parola. Capisco che a una certo punto si arriva al voto, ma quando avevo alzato la mano non si era ancora in fase di votazione. Voglio dire sommessamente al collega Nitto Palma che abbiamo letto quel testo normativo, lo conosciamo e ne abbiamo visto le diverse sfaccettature. Esso, da un lato, stabilisce che il diritto al soggiorno possa venire in meno in quanto lo straniero in Italia non abbia fonti di reddito, sia cioè nullatenente; quindi, dopo i primi tre mesi di soggiorno può può esservi un accertamento del prefetto e una valutazione sulla sua condizione. Ma intanto, collega Nitto Palma, ella non potrà non ammettere, avendo letto la norma, che questa previsione non è automatica, che non vi è cioè un automatismo tra l'assenza di fonti certe di sostentamento e il provvedimento di espulsione. In questo senso la direttiva europea è molto chiara ed è altrettanto chiaro il decreto legislativo n. 30 del 2007. Se si ritiene che questa norma debba essere corretta in senso più restrittivo, tale correzione non può che passare attraverso una concertazione tra i Paesi dell'Unione e una nuova direttiva che indichi criteri più restrittivi. In questo momento la legge italiana non può introdurre criteri più restrittivi rispetto a quelli della direttiva recepiti nel decreto legislativo

la direttiva europea parla chiaro: essa stabilisce che occorre fissare un termine non discriminatorio e congruo. Ma la fissazione di questo termine non discriminatorio e congruo, lei sostiene, non può essere effettuata se non con una norma di legge. Su questo ho un dubbio e mi permetto di dissentire.

termini che corrispondano a tale criterio? Credo di sì. Il criterio è fissato legislativamente, esso deriva da una direttiva europea che necessariamente deve avere un carattere generale e deve fissare un criterio generale. Dopodiché, arriva il provvedimento del Ministro e questo può definire dettagliatamente le modalità di applicazione di quel criterio. il termine fissato attraverso il provvedimento del Ministro non è congruo ed è discriminatorio, naturalmente ciò potrà essere valutato ed accertato in sede di ricorso contro il provvedimento di allontanamento. A me sembra che le motivazioni fondamentali alla base delle tesi che sono state qui sostenute da esponenti illustri dell'opposizione siano complessivamente poco rilevanti e, anzi, destituite di fondamento. Per questa ragione, credo che il subemendamento in discussione debba essere respinto e ritengo sia invece più corretto più coerente con il decreto‑legge nel suo insieme e con la normativa europea procedere, appena possibile, all'approvazione dell'emendamento 1.300, presentato dal Governo.

del professor Brutti di sostenere con tanta consequenzialità logica l'esatto contrario di quanto è scritto nella direttiva. Il Governo, nel momento in cui ha recepito la direttiva,

Ha cambiato alcuni termini - e da ciò la necessità, nel decreto-legge, di spostare sul prefetto le competenze che erano state attribuite esclusivamente al Ministro dell'interno - e ha ritenuto di non recepire il comma 5 dell'articolo 5 della direttiva. Signor Presidente, il comma 5 dell'articolo 5 prescinde, a differenza di ciò che ha detto poco fa il senatore Brutti, da qualsiasi questione relativa al reddito. Vorrei capire come si faccia a stabilire in modo certo l'adempimento di un obbligo se non si fissa un termine altrettanto certo per adempierlo. È una norma garantista che punta ad avere certezza e chiarezza in questo testo di legge.

fra l'altro dedica una grande attenzione (i fatti di ieri lo dimostrano in maniera importante e positiva): l'opera delle Forze dell'ordine e della magistratura in Sicilia. Ho presentato la citata interrogazione per il potenziamento delle Forze dell'ordine nella stazione dei Carabinieri di Zafferana Etnea, con atto pubblicato nella seduta n. 167 del 13 giugno 2007. Non ho ancora, a distanza di quattro mesi, ricevuto risposta;